La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato il calendario dei lavori fino al 16 febbraio. Nella seduta di oggi sarà discusso il decreto-legge recante interventi urgenti per la popolazione di Ischia, approvato dalla Camera dei deputati. La seduta di domani avrà inizio alle ore 10,30 con il ricordo del Giorno della memoria. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti. L'ordine del giorno della seduta di domani prevede inoltre il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time* con la presenza dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura e della sovranità alimentare e del lavoro e delle politiche sociali. Il calendario della prossima settimana prevede i seguenti argomenti: deliberazioni sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge in materia di introduzione del reato di omicidio nautico e per cinque ratifiche di accordi internazionali; disegno di legge di ratifica degli Accordi Italia-Svizzera su lavori frontalieri e doppie imposizioni; dalla sede redigente, disegno di legge istitutivo di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; riforma del Regolamento del Senato recante introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura, per il quale è previsto il voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Giovedì 2 febbraio si svolgeranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time* con la presenza dei Ministri della difesa, della salute e dell'università e della ricerca. L'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 6 al 10 febbraio, in vista delle elezioni regionali previste per domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Le Commissioni potranno convocarsi in relazione a esigenze dei rispettivi programmi dei lavori. Il calendario della settimana dal 14 al 16 febbraio prevede la discussione dei seguenti argomenti: decreto-legge proroga termini; dalla sede redigente, disegno di legge recante introduzione del reato di omicidio nautico, per il quale sia stata accolta la procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento; ratifiche di accordi internazionali per le quali sia stata accolta la procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Giovedì 16 febbraio si svolgeranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

*relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono passati poco più di due mesi da quando, quel tragico 26 novembre 2022, colate di detriti e fiumi di fango hanno distrutto abitazioni e attività e causato dodici vittime. Il dolore e lo sgomento per quanto accaduto a Ischia sono ancora presenti più che mai dentro tutti noi. Ecco perché anche oggi in questa sede, mentre ci confrontiamo sull'esame del decreto-legge e sugli interventi che daremo alla popolazione colpita da quei movimenti gravitativi distruttivi, è quanto mai doveroso rivolgere un pensiero commosso e partecipe a tutte le famiglie colpite, ai congiunti delle vittime e a quanti soffrono le conseguenze di questa tragedia. Allo stesso modo, cogliamo l'occasione per ribadire tutto il nostro apprezzamento e la più sentita gratitudine alle donne e agli uomini che sono accorsi in aiuto della popolazione: dai Vigili del fuoco, alle Forze dell'ordine, ai sanitari, al mondo del volontariato e soprattutto alla Protezione civile. È stato grazie al loro tempestivo intervento se oggi facciamo un bilancio meno grave. D'altra parte, è importante riflettere sul valore della prevenzione, della programmazione e della sostenibilità degli interventi dell'uomo sulla natura e sui paesaggi. La coscienza della fragilità della natura idrogeologica del nostro Paese, in contrasto all'organizzazione selvaggia e senza criterio, è la base necessaria per evitare in futuro nuove tragedie come quelle di Ischia. Il progresso e il rispetto dell'ecosistema e la messa in sicurezza del territorio non sono elementi tra loro antitetici; anzi, esistono metodi e tecnologie innovative che riescono a contemperare e a rafforzare il legame tra queste irrinunciabili esigenze. Si tratta di un percorso e di un obiettivo che questo Governo ha ben chiari e che mi auguro possano trovare le più ampie convergenze politiche in entrambi i rami del Parlamento. Lo dobbiamo a chi ha perso tutto. Lo dobbiamo alle generazioni future. Come è noto, il Governo e, subito dopo, il Parlamento hanno immediatamente agito per fronteggiare l'emergenza, attraverso lo stanziamento e l'erogazione di appositi fondi. Ora, terminata la prima fase, si tratta di dare forza e continuità alle misure messe in atto per sostenere anche nel futuro la popolazione colpita. Voglio ricordare che il 27 novembre il Consiglio dei ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza e stanziato 2 milioni di euro sul Fondo per le emergenze nazionali per

Il documento oggetto del nostro confronto è già passato all'esame della Camera dei deputati e nel corso dei procedimenti si è arricchito di nuovi e importanti elementi. Innanzitutto, a favore dei soggetti aventi la residenza ovvero la sede legale operativa nei Comuni i commi da 1 a 4 dell'articolo 1 dispongono la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Ai sensi del comma 5, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazioni di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2023. Il comma 6 prevede che, per i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applica la disciplina in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali. Il comma 7, allo scopo di assicurare ai Comuni interessati il gettito dei tributi non versati, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1,340 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,380 milioni per l'anno 2023. L'articolo 2 detta disposizioni in materia di giustizia civile e penale disponendo, in primo luogo, il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia. Nei medesimi procedimenti dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Il rinvio delle udienze è disposto anche, su istanza di parte, nei procedimenti pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari in cui vi siano parti o difensori residenti o che svolgano la propria attività alla data del 26 novembre 2022 nei Comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Inoltre, si prevede nei confronti dei soggetti residenti o che svolgono la propria attività nei predetti Comuni alla medesima data del 26 novembre 2022 la sospensione dei termini perentori, legali o convenzionali, per l'esercizio di azioni o del diritto alla presentazione di ricorsi. Il comma 6 elenca i casi in cui le disposizioni predette non trovano applicazione. L'articolo 3 dispone la sospensione dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 dei termini processuali nell'ambito di giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno. Nei suddetti giudizi le udienze fissate nel medesimo arco temporale sono rinviate su istanza di parte a data successiva. L'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia. L'articolo 5 destina 10 milioni di euro per l'anno 2022 al Fondo regionale di protezione civile. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono stati inseriti gli articoli da L'articolo 5-*bis* autorizza l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale a reclutare a tempo indeterminato fino a 90 unità di personale per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico, un intervento - a mio avviso - fondamentale. L'articolo 5-*ter* attribuisce al Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, anche i compiti relativi agli interventi riferiti agli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 regolati dall'articolo in esame e prevede che il Commissario straordinario predisponga un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre, che contiene anche una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia. Il piano ha validità quinquennale ed è approvato con ordinanza commissariale, acquisito di parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e sentita la Regione Campania. Per gli interventi di conto capitale è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. L'articolo 5-*quater* prevede che l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale aggiorni gli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia che - ribadisco - Sono disciplinate altresì le modalità dell'aggiornamento del piano su più stralci funzionali. l'applicazione delle semplificazioni per l'affidamento dei contratti sotto soglia previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020. L'articolo 5-*sexies* attribuisce al Commissario straordinario il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti relative alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata

la dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di 3,61 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028. I commi 2 e 3 dispongono la norma di copertura finanziaria Grazie a tutti nelle giornate passate, mi auguro che anche in questa occasione il confronto e la dialettica si possano sviluppare attraverso un clima di serena discussione e collaborazione tra tra tutti noi, tra le forze di maggioranza e opposizione, nell'esclusivo interesse della gente di Ischia, per giungere a un risultato che ci veda convergenti e che possa dare risposte vere e concrete a tutta la popolazione. *(Applausi)*.

Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, cosa si può dire di più davanti a un'immane tragedia come quella di Ischia, una tragedia che si è portata via la vita di intere famiglie? Poteva accadere anche a me, mentre dormivo sicuro nella mia abitazione. Le ultime immagini trasmesse quarantotto ore fa dalla stampa locale riprendono via Pennino, strada di Casamicciola Terme, inondata da un fiume di acqua e fango. fango. La parola "emergenza" richiama un concetto legato a una circostanza imprevista recante un'accezione temporalmente circoscritta. Ma, se a ogni pioggia il Commissario competente evacua centinaia di abitanti, si può parlare di emergenza? A me sembra che l'abuso di questo termine sia un po' un paravento dietro cui nascondere le parole "programmare", "pianificare" e "prevenire". Come sarebbe bello se in questo Paese potessimo abusare di più della parola "prevenzione" invece che della parola "emergenza". Prevenzione vuol dire fare interventi strutturali e l'isola di Ischia - come abbiamo sentito - ha bisogno di interventi strutturali. quest'isola è stata sconvolta da numerosi eventi, da terremoti e frane anche in anni passati, che hanno ucciso - l'avete ricordato in quest'Aula - nel 1883 2.300 persone, la famiglia di Benedetto Croce. Eppure, il sommo letterato non descrisse l'isola come un paradiso abitato da diavoli. Croce non si sarebbe mai sognato di attribuire agli stessi isolani la tragedia di un'isola che tanto fu cara a Montale e Morante. Ma qui c'è il pregiudizio verso il Sud tipico di una parte della politica e di tanti partiti che hanno il loro *leader* al Nord e di alcune testate giornalistiche che hanno editorialisti poco onesti intellettualmente. Certa stampa nazionale, riesumando riesumando le teorie lombrosiane, ha ricondotto la catastrofe del 22 novembre alla mano umana, mentre le alluvioni che accadono in altri paesi di altre parti d'Italia continuano a a dipendere esclusivamente dai cambiamenti climatici. È la solita discriminazione di una parte di questo Paese, il solito *cliché*, e così al fango si è aggiunto altro fango. E in quel fango ha sguazzato anche il senatore Renzi, giusto per l'ossessione che ha per il MoVimento 5 Stelle e per Giuseppe Conte. *(Applausi)*. Ma dobbiamo concentrarci tutti, in quest'Aula, sul fango dei politici o sulle centinaia di nostri concittadini che stanno dormendo in case di amici, familiari, arrangiandosi in alberghi? Io non ho dubbi rispetto a chi dobbiamo concentrarci e a chi dobbiamo prestare attenzione. Quegli uomini e quelle donne meritano una risposta alle domande: domani dove dormirò? Domani dove costruirò la mia casa? Dov'è la risposta in questo decreto? Relativamente, poi, ai fondi messi a disposizione, di cui abbiamo sentito, io non posso stabilire se siano adeguati. Ma certamente mi posso rimettere alle parole dei sindaci dell'isola, come il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, che ha testualmente riferito che gli stanziamenti messi a disposizione potrebbero, al massimo, servire per ripulire il fango. E chi più di un primo cittadino ha il polso della situazione? Inoltre, mi chiedo perché in simili altre parti del Paese i familiari delle vittime hanno avuto accesso a un fondo speciale, contrariamente a quanto avvenuto per l'isola di Ischia. Penso alla catastrofe di Rigopiano, dove è stato corrisposto un importo di 200.000 euro a ciascun familiare delle vittime. Gli ischitani, quindi, per questo Governo sono considerati cittadini di serie B? Il commissario Legnini, il cui operato è apprezzato dalla comunità isolana, necessita di norme chiare, precise ed esaustive, così come ha bisogno degli stessi uomini e stanziamenti messi a disposizione per eventi analoghi. Onorevoli colleghi, un Governo serio si sarebbe prodigato per assicurare una pulizia degli alberi e dei pendii, un ripristino immediato delle opere idrauliche e dei sentieri, seri interventi di monitoraggio, uno studio volto ad analizzare tutte le opere e la staticità degli immobili. Invece, niente in questo decreto. richieste, queste ultime, avanzate anche da una attivista del MoVimento 5 Stelle di Casamicciola, l'architetto Caterina Iacono; richieste ancora una volta inascoltate. Finito di piangere le vittime, il problema viene rimosso, fino alla prossima tragedia. Perciò, non da senatore della Repubblica, ma da figlio di questa terra, chiedo ed esigo dal Governo che venga predisposto in tempi certi un piano per la difesa del suolo, uno studio sul dissesto idrogeologico dell'isola capace di mettere in rilievo tutte le aree soggette a frane, a rischio sismico alluvionale e a rischio di rottura della superficie. Poi, c'è un altro capitolo che dobbiamo aprire, che è quello del personale amministrativo dell'isola, che andrebbe incrementato. È impensabile, infatti, che in queste amministrazioni i funzionari preposti al rilascio della carta d'identità poi si debbano occupare delle pratiche della ricostruzione. Così si blocca tutto.

di ricostruzione. Evidenzio la parola isola. Come già richiesto dai sindaci, questo decreto avrebbe dovuto interessare l'intera isola, ma non si è fatto. Onorevoli colleghi della maggioranza, mi chiedo e vi chiedo: ma voi le audizioni dei soggetti direttamente interessati le avete ascoltate? Confrontando questo decreto con le richieste avanzate dai sindaci del territorio di Ischia - del territorio e non dei Comuni di Ischia - io resto basito innanzi all'insensibilità di chi si è curato solo di accendere i microfoni dei primi cittadini ischitani in Commissione, quasi che fosse un atto dovuto, non curandosi di dar seguito alle loro più legittime richieste. Personalmente, ritengo una mancanza di rispetto invitare i sindaci nelle Commissioni parlamentari e limitarsi a offrire loro il caffè, facendo finta di prendere appunti, salvo poi disattendere la stragrande maggioranza delle loro richieste. Per questo io, che quelle audizioni le ho seguite da remoto, non facendo parte delle Commissioni competenti, non posso che fare mie le parole pronunciate da Giacomo Pascale: Ischia, fra non molto, dovrà attrezzarsi per la nuova stagione turistica dovranno abbracciare decine di migliaia di turisti in totale sicurezza. L'auspicio è che questa emergenza non finisca mai, a questo punto, nel senso che occorre mettere in sicurezza, una volta e per tutte, il territorio,

un Paese dove spesso il potere mediatico detiene le redini del potere politico. Non si abbassi, dunque, la guardia. Sostituiamo finalmente alla parola «emergenza» la parola «prevenzione».

e dai prossimi provvedimenti. Il MoVimento 5 Stelle c'è, con il suo impegno. Stiamo però aspettando i voti della maggioranza - lo ripeto - sulle nostre proposte emendative che non sono state ascoltate e rispetto alla voce inascoltata dei sindaci. sindaci. Termino il mio intervento con una frase di Victor Hugo: forse, grazie all'interessamento di tutti, questa volta finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole.

tragedie come quella successa a Ischia il 26 novembre scorso hanno il potere di fermare il tempo e, peggio, di portare indietro le lancette. A Ischia il dramma del 2022 si accoda a quello del 2017:

la sua evoluzione naturale, non si cura dei nostri affanni e del nostro dolore per le tragedie accadute. Noi, però, abbiamo gli strumenti: l'ingegno, la tecnica, il progetto.

La storia insegna: nel passato ci siamo sempre difesi con ripari, con fortificazioni, con ogni conoscenza tecnica che avevamo a disposizione. Ora dipende da noi, dal nostro impegno, dal senso di responsabilità voler mettere in sicurezza il territorio. Dobbiamo difenderci meglio, ma finora non lo abbiamo fatto: abbiamo fatto sempre e solo annunci. parlato della prevenzione, ma mi risulta che anche il Governo con i 5 Stelle ha addirittura smantellato la struttura di missione "Italia sicura" e "Casa Italia", a cui erano stati assegnati dei finanziamenti

lo Stato ha il dovere di aiutarlo a ricominciare. Da una parte, ci sono le esigenze di vita quotidiana dei cittadini del luogo; dall'altra, c'è una prima forma di interventi tampone per mettere in sicurezza lo stato dei luoghi, con la previsione di un Commissario straordinario, in attesa di un piano complessivo che riguardi i rischi idrogeologici dei quali il nostro Paese è specificatamente connotato. La vita di un territorio così colpito ha la necessità di fermare alcune fasi della propria quotidianità. Nell'immediato era necessario disporre la sospensione di una serie di termini, di versamenti e di adempimenti tributari e contributivi, nonché di rinviare le udienze di procedimenti civili e penali. Si è pensato anche a sostenere i Comuni interessati che hanno perso il gettito dei tributi sospesi, prevedendo un apposito fondo tenuto presso il Ministero dell'interno. All'Italia, però, serve un progetto complessivo di salvaguardia del territorio sul piano idrogeologico, energetico e sismico. Abbiamo le competenze per poterlo fare. Abbiamo i tecnici e abbiamo le imprese. D'altra parte, già l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha fatto comprendere che, oltre alle misure immediate, fosse necessario rendere ancora più concreti gli interventi economici. Si è arrivati infatti a stanziare fino a 85 milioni di euro. Le modifiche alla Camera hanno ulteriormente ampliato il raggio di azione del decreto, prevedendo il rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. Al Commissario straordinario, nel 2017, sono stati anche assegnati i compiti relativi agli interventi del novembre 2022. Questo è logico, oltre che assolutamente necessario, per garantire il coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e quelli di ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili privati. Così come è fondamentale avere una visione pluriennale per la ricostruzione, il Commissario ha anche il compito di predisporre un piano di interventi con una validità quinquennale. Sempre per pianificare gli interventi, è stato previsto che l'Autorità di bacino si occupi dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione. Ciò è importante perché può avvenire poi per più stralci funzionali. Se però è apprezzabile questa emergenziale ed embrionale prima forma di tutela delle persone e del territorio, la discussione deve essere anche l'occasione per un ripensamento complessivo del ruolo del Governo, statale, regionale e locale, riguardante un problema atavico che la nostra terra, bellissima e meravigliosa, ha nel suo bagaglio. La cura di un'Italia tanto bella, ma tanto delicata per la sua connotazione idrogeologica, merita un approccio che non può essere solo di tipo emergenziale e successivo alle tragedie. L'abusivismo è un dato di fatto incontestabile, un problema su cui si deve intervenire in maniera decisa e soprattutto netta. È

per il rischio idrogeologico. Urge quindi un programma di monitoraggio più costante e analitico delle aree più a rischio. Ecco perché è importante l'ordine del giorno sull'unità di missione per il monitoraggio e il coordinamento del dissesto idrogeologico. Si potrebbe anche in qualche modo collegare questa unità di missione alle Agenzie regionali per la gestire da remoto sia il monitoraggio che un programma di dati utile sia per l'emergenza che per la previsione di progetti di prevenzione. non basta. Per il futuro sarebbe anche opportuno pensare a un codice dell'emergenza, che si attivi *ipso iure* in caso di calamità idrogeologica, prevedendo un ampio ventaglio di tutele e accorgimenti nel caso di evento infausto. Non può e non deve essere il Governo di turno a decidere se vanno sospesi i processi, le rate dei mutui o i tributi. L'esperienza, purtroppo negativa, sulla tematica in questione ci ha insegnato quali possono essere le più opportune misure in casi di questo tipo. Sarebbe opportuno quindi pensare a una legislazione più complessiva

dovere è garantire sicurezza alle persone e salvaguardare un patrimonio unico al mondo. Oggi non abbiamo alibi, ce lo chiedono i sopravvissuti, lo impone la storia. Serve un grande programma nazionale di investimenti e incentivi, un'operazione di sistema che deve partire subito e che ha bisogno di tempi lunghi. D'altra parte, la natura ragiona su tempi molto lunghi. È quindi importante avviare un grande progetto complessivo, sul serio questa volta. Il nostro territorio va salvaguardato e difeso; ce lo chiedono da anni proprio eventi del genere. La straordinaria bellezza dei nostri luoghi è un valore profondo. L'obiettivo a cui dobbiamo aspirare, dopo le disgrazie avvenute e i tanti morti, è una grande operazione di salvaguardia per il futuro, rifiutare l'alibi della fatalità, difendere le vite umane e proteggere questa nostra grande bellezza. Questo è il nostro compito di legislatori.

travolge e porta via tutto il fango, scendendo dalla parte alta di via Celario e arrivando giù, fino a piazzale Anna De Felice; già, una frana disastrosa che si riversa su un piazzale che porta il nome di una vittima di una frana disastrosa. Aveva quindici anni Anna De Felice nel 2009. Ischia: breve cronistoria di un evento nefasto. Ebbene, Presidente, è in momenti come questi che bisognerebbe concentrare tutte le nostre energie su elementi fondamentali, elementi importanti per una programmazione corretta, seria ed efficace, che non può prescindere dal dove, dal come e dal quando. Signor Presidente, Ischia non si sottrae all'infausta statistica che vede il 94 per cento dei Comuni italiani a rischio di dissesto idrogeologico. Ischia rappresenta un'istantanea del nostro Paese. E l'immagine che ci ritorna racconta di disastri annunciati e morte; di territori vocati, per tradizione e storia, alla bellezza e al benessere, ridotti in cumuli di macerie che, nel loro percorso di devastazione, strappano alla vita anime innocenti. Dunque, Presidente, il dove è rappresentato dall'insieme dei luoghi che necessitano di misure per la mitigazione del rischio idrogeologico, individuabile tramite la carta geologica d'Italia, e dal progetto Carg, che al momento, però - Presidente - grazie alle esigue risorse messe a disposizione da questo Governo, fornisce solo una copertura al 50 per cento del Paese. Mancano ancora 335 fogli per il completamento del restante 50 e non certo con strutture sottodimensionate come "Italia sicura". Dunque, Presidente, diventa evidente che non si può prescindere dalla conoscenza del territorio come elemento fondamentale per la prevenzione e la messa in sicurezza. E come pensiamo di farlo se si taglia il 40 per cento delle risorse per il dissesto idrogeologico? Direte che i soldi mancano, ma 900 milioni per le squadre di calcio si trovano e, chissà, magari anche di più, con il beneficio fiscale del rimpatrio dei cervelli, esteso anche ai rinnovi contrattuali calcistici. Negli ultimi tredici anni in Italia si sono susseguiti circa 1.500 eventi calamitosi, da Nord a Sud. Eppure, da dieci anni si discute di una legge che vieti il consumo di suolo. Ischia, Presidente, al pari degli altri siti interessati, negli ultimi anni chiede e necessita di un supporto economico che ridia dignità a una popolazione profondamente ferita. I sindaci dell'isola verde - la cui maggioranza è identificabile con le forze di centrodestra - hanno chiesto un fabbisogno di 400 milioni. Con questo decreto-legge ne viene concesso appena il 10 per cento, con il quale a stento si potranno rimuovere i detriti e, probabilmente, si pulirà il piazzale dedicato ad Anna De Felice, spazzato via dalla colata di fango di novembre. Il come è rappresentato dal combinato disposto delle misure per la mitigazione del rischio idrogeologico e il contrasto serrato agli abusi edilizi, su cui negli anni nulla è stato fatto e su cui alcuni membri di quest'Assemblea hanno speculato, accreditando a questa forza politica un condono edilizio mai esistito. Anzi, cito è impossibile pensare di fare decine di migliaia di demolizioni, si rischia di creare un problema abitativo. Sono le parole di Giosi Ferrandino, per dieci anni sindaco di Casamicciola, e altrettanti anni sindaco di Ischia, attuale europarlamentare di Italia Viva, che nel 2012 fece un'alleanza alle elezioni amministrative con il centrodestra per la difesa di 700 immobili abusivi, destinatari di 700 decreti esecutivi di abbattimento. È evidente, Presidente, che le risorse messe in campo sono insufficienti e le azioni perentorie inesistenti, e, nonostante si chieda una partecipazione trasversale, a cui il MoVimento 5 Stelle, certo, non si sottrae, tengo a evidenziare che i nostri emendamenti, richiesti dai sindaci dell'isola, non sono stati approvati. In merito al quando, Presidente, sembra pleonastico dire che la tempistica degli interventi non è più procrastinabile: il quando non può essere che ora. il giudizio sul provvedimento in esame non può che essere positivo. L'isola di Ischia e i Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno avevano bisogno di una risposta, che è arrivata. Si tratta naturalmente di un primo passo, che tiene conto delle esigenze raccolte attraverso molte audizioni e un confronto propositivo con tutte le istituzioni territoriali. Prima di entrare nel merito del testo in esame, sia permesso al nostro Gruppo parlamentare di rimarcare come anche questa tragedia sia avvenuta pur esistendo una precisa cognizione del frangente di rischio. Le più recenti informazioni note - come quella, ad esempio, contenuta nel rapporto sul dissesto idrogeologico del 2021, targato indicano l'esatta quantificazione dei cittadini e delle famiglie esposte a un rischio idrogeologico, indicando "dove", "come" e forse, per qualche situazione, non è del tutto escluso poter dire anche "quando". Di certo, a ogni evento atmosferico di maggiore entità, almeno 548.000 sono le famiglie a rischio per frane e sono 565.000 gli edifici a rischio di eventi calamitosi, poiché ubicati in aree inondabili. La stessa Regione Campania ha stimato che il 49 per cento del territorio di Ischia è da considerare a pericolosità elevata. Ebbene, ritengo che per queste aree non possiamo più confondere la mera condizione di regolarità amministrativa come un sinonimo di sicurezza abitativa. È evidente come nel nostro Paese non possa più considerarsi valida una coincidenza tra regolarità dei titoli abilitativi, magari rilasciati sulla base di criteri e di norme di oltre cinquanta o sessanta anni fa, e la non pericolosità del territorio. Continuare a ripararsi dietro questo debole appiglio corrisponde all'evidente volontà di rifiutare una diretta rispondenza tra il mutevole stato di pericolosità dei luoghi e i nuovi fenomeni climatici. Inoltre, significherebbe rifiutare gli effetti migliorativi derivanti dalla sicurezza normativa che, grazie alle ultime novità introdotte anche recentemente in ambito normativo, vede i cittadini maggiormente tutelati dagli stringenti dettami normativi sorti dopo tragedie come quella, ad esempio, di Sarno. È bene essere chiari: spesso ci preoccupiamo del rispetto delle formalità richieste dalle norme in vigore, realizzando magari azioni a macchia di leopardo di ordinaria e straordinaria manutenzione, ma non certamente di prevenire, attraverso un'operazione organica, disastri annunciati. Anche per la carenza di risorse ci si arrende ad aspettare passivamente la prossima emergenza. Quello di Ischia non è purtroppo un episodio limitato, ma è uno degli eventi ciclici che periodicamente dobbiamo mettere in conto che si ripetano con uguale intensità. Basta con i messaggi distorsivi post-tragedia! Abusivismo, cambiamento climatico, zone di rischio note che non hanno originato regole vincolistiche, totale o carente manutenzione del territorio: sono molte le ritenute concause, individuate sin dalle prime ore successive al disastroso evento che ha colpito l'area dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, sull'isola di Ischia. La verità è forse che, sino alle ultime ore prima dell'evento, le peculiari e meravigliose caratteristiche storiche, paesaggistiche e climatiche del territorio nazionale ci hanno illuso e ci illudono che quelle stesse meraviglie geo-ambientali, in cui la maggior parte della popolazione italiana si trova ad abitare, siano estranee alle azioni del clima e della natura. Citerò per tutte la tragedia di Rigopiano, a significare quanto imprevista e ineluttabile sia l'azione naturale dei fenomeni, allorché venga del tutto ignorato il rispetto di basilari regole di precauzione e ci si muova purtroppo, in funzione di prevalenti utilità economiche. È così che oggi, in questa sede parlamentare, dopo aver pianto la scomparsa delle vittime della tragedia, ci troviamo a convertire in legge il decreto-legge recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola Il testo normativo disciplina - come detto - i primi interventi urgenti in favore delle popolazioni interessate, colpite da eventi alluvionali franosi di eccezionale intensità, che hanno provocato morti, una grave situazione di pericolo per le persone e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Le misure sono volte essenzialmente a disciplinare la sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali, anche su istanza di coloro i quali - ad esempio difensori o parti processuali residenti nei Comuni interessati dall'evento siano parte di processi pendenti in sedi diverse da quelle della sezione distaccata del tribunale di Ischia che ha avuto, con lungimiranza, una proroga del termine di sopravvivenza che, altrimenti, sarebbe stato quello del 31 Nel corso dell'esame in sede referente è da lodare un'iniziativa che ha permesso di apportare diverse integrazioni. Sono stati attribuiti al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma a Ischia nel 2017 anche i compiti relativi agli interventi riferiti agli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, al fine di garantire il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e il ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili privati a seguito degli eventi calamitosi di cui ci stiamo occupando. Viene prevista la predisposizione di un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre ed è prevista la spesa di circa 40 milioni di euro per il periodo 2023-2026. Ulteriori disposizioni introdotte in sede referente prevedono l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia e disciplinano le procedure finalizzate all'affidamento dei servizi di progettazione ed dei lavori relativi agli interventi individuati nel piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia, incrementando naturalmente le unità di personale della struttura a supporto del Commissario.

sono di fatto ancora in pericolo. È compito del legislatore e di questa maggioranza dedicare alla sicurezza della comunità ogni e più ampia attenzione. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a convertire in legge il decreto-legge recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre, approvato non senza difficoltà e polemiche la scorsa settimana dei deputati. Le misure contenute nel decreto-legge spaziano dalla sospensione di alcuni adempimenti tributari al rinvio delle udienze civili e penali, passando per l'aumento delle risorse destinate al fondo di Protezione civile; un piano commissariale per Ischia che aiuti a superare la compromissione degli interessi primari della popolazione; un piano atteso, sin qui mai realizzato, per il contrasto al dissesto idrogeologico dell'isola, benché la necessaria predisposizione fosse prevista anche per la ricostruzione post-sisma. Questo decreto-legge è purtroppo l'emblema di un modo sbagliato di governare il nostro Paese ormai da lunghissimi anni, in uno dei settori più importanti per il futuro, ovvero la cura del territorio e la prevenzione dei rischi legati al dissesto idrogeologico; un fenomeno quest'ultimo che, al di là delle cause che possono averlo generato (lo spontaneismo edilizio, l'assenza di pianificazione urbanistica, finanche i bisogni della vita), non ammette scuse e va condannato senza appello. Lo Stato è colpevole nei confronti dei suoi cittadini quando aspetta il verificarsi di un evento estremo o di una vera e propria tragedia, così come purtroppo è stata quella che si è verificata a Ischia tra il 25 e il 26 novembre 2022. Insomma, la logica dovrebbe essere esattamente il contrario, e cioè prevenire. Prevenzione infatti dovrebbe essere la parola chiave con la quale iniziare ad affrontare la questione. Prevenzione, inoltre, è anche la parola chiave che servirebbe davvero per risparmiare le risorse, anche fino all'80 per cento di tutto ciò che si spende, continuando a inseguire le emergenze, per riparare i danni. Invece, ancora una volta, frane e allagamenti hanno causato l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni: 1.500 sfollati, che si aggiungono a quelli del terremoto; danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e agli edifici pubblici e privati; nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione. Drammatico è il bilancio delle vite umane: dodici persone sono decedute, tra cui quattro bambini. I tempi che la legge ci concede per poter convertire in legge questo decreto-legge sono brevissimi (entro il 1° febbraio). colleghi, che gli elementi per avere un quadro chiaro della situazione di rischio che vive l'isola ci sono tutti e da molto tempo. Eppure, nel corso degli anni le azioni concrete di prevenzione sono state praticamente nulle. Questa nuova tragedia ci obbliga a ricordare come il nostro sia un Paese fragile, segnato dal dissesto idrogeologico, da un consumo di suolo dissennato e dall'abusivismo edilizio. Questa, dunque, poteva essere, da parte del Governo, l'occasione per iniziare un percorso diverso, in grado di uscire dalla prospettiva inaccettabile di inseguire le emergenze, provando a tamponare ogni qualvolta si verifica una tragedia, e mettere in campo invece una strategia compiuta di prevenzione e cura del territorio, che avesse una visione di come cambiare passo e mettere in sicurezza l'isola, una visione che andasse più in là nel tempo. Il decreto-legge, da questo punto di vista, è del tutto insufficiente e, solo grazie agli interventi emendativi arrivati dal Partito Democratico, è stato possibile renderlo quantomeno più adeguato alle esigenze dei Comuni interessati dagli ultimi terribili eventi atmosferici. Mancavano e mancano ancora le risorse necessarie a garantire interventi concreti, finalizzati alla messa in sicurezza del territorio dell'isola di Ischia. Non possiamo certo dire che si tratta di un evento che coglie di sorpresa né le amministrazioni locali, né il Governo nazionale. In Italia i disastri ambientali, come la strage di Ischia, sono figli del *modus operandi* che si registra ogni qualvolta avviene una tragedia. Come sempre capita nel nostro Paese, la tragedia si raddoppia: dopo la valanga di fango c'è quella della demagogia, delle chiacchiere al vento. Dopo il terremoto del 2017 a Ischia o le alluvioni, come quella nelle Marche, hanno fatto seguito la ricerca dello scandalo, le accuse su chi non ha fatto cosa, soldi non spesi, senza alcuno sforzo per capire le ragioni del disastro, le cause dei ritardi, i problemi veri. La fragilità del territorio dell'isola era quindi nota da tempo. Questo, però, non è stato sufficiente per un reale risveglio delle coscienze e una riforma organica della gestione e della manutenzione del territorio, in grado di mettere in sicurezza quell'isola: le sue abitazioni, la vita dei cittadini e le reali e concrete possibilità di sviluppo turistico, indissolubilmente legate alla salvaguardia di ambiente e territorio e alla sua sicurezza. Proseguire invece lungo questa strada vuol dire dare il via libera alla prassi alla quale abbiamo assistito: una letale combinazione tra malagestione del territorio ed eventi climatici estremi, che si fanno sempre più frequenti e drammatici, anche in relazione ai cambiamenti climatici ai quali siamo assistendo, senza aprire un dibattito franco, aperto e complessivo sul modo con il quale affrontarli. Uno dei punti fermi dai quali partire - e quanto verificatosi ad Ischia lo dimostra una volta di più - è rappresentato dalla lotta all'abusivismo, che si può vincere soltanto con una logica di rigore estremo. Avete detto «no» alle proposte del PD che volevano evitare che questo decreto-legge rimanesse uno strumento vuoto e privo delle risposte che i cittadini di Ischia aspettano da lungo tempo. Le amministrazioni locali non possono essere lasciate da sole e per questo, senza essere ascoltati, abbiamo a lungo insistito sulla necessità di sostenere le amministrazioni locali rispetto alle difficoltà che avranno a ripagare i mutui con il MEF e per i mancati introiti legati alla Tari, che ovviamente non riceveranno nei prossimi mesi. Abbiamo chiesto di aiutare le famiglie, chiedendo di non far pagare l'Imu a quelle che non saranno più nella possibilità di abitare i loro edifici. È irragionevole chiedere di pagare l'Imu su un'abitazione inagibile. Purtroppo, su questi punti abbiamo trovato un Governo che non ha voluto prestare ascolto. L'Esecutivo deve dirci con chiarezza se vuole aiutare o meno le comunità interessate dagli eventi calamitosi, e non può certo pensare di svicolare nascondendosi dietro raccomandazioni fumose. Lo stanziamento di 40 milioni di euro in quattro anni, stabilito dal decreto-legge risulta esiguo e non corrispondente alle richieste del Commissario per l'emergenza. Come è stato più volte ribadito nel corso dell'esame parlamentare, questo decreto-legge, giudicando le risorse introdotte, è comunque insoddisfacente e parziale. Ci aspettiamo che dopo questa tragedia si apra una riflessione generale sulle questioni legate alla prevenzione dal dissesto idrogeologico, alla cura del territorio, alle modalità più congrue ad affrontare i cambiamenti climatici in atto. Mi preme però sottolineare

per gli appalti pubblici, in esame alle Commissioni ambiente di Camera e Senato, in cui sparisce la compatibilità geologica e idrogeologica del territorio. *(Applausi)*. Ho ascoltato con grande rispetto alcune relazioni dei colleghi di maggioranza che dicono: bene il decreto, ma dobbiamo fare un piano sulla prevenzione, dobbiamo fare degli interventi strutturali. Allora non diciamolo solamente, facciamolo. La prima prova sarà quella di riformare la proposta sul nuovo codice degli appalti, che invece attualmente nell'idea di semplificare ha eliminato la compatibilità geologica e idrogeologica.

la mia sarà forse una voce controvento. Ma, nonostante tutto,

leale confronto, condivisione e responsabilità rispetto al dramma che ha vissuto e sta vivendo la comunità di Ischia; un dramma che ho avvertito in tutte le parole dei senatori che hanno preso la parola e il cui contenuto ho profondamente condiviso nel merito. Un diplomatico, uno dei protagonisti della Terza Repubblica francese, parlando proprio di Ischia, ebbe a dire che il sole radioso di quel tratto di cielo riusciva a trasfigurare ogni cosa, anche la morte. Ebbene, credo che il modo migliore che ha quest'Assemblea e ciascuno di noi per onorare la morte, per onorare le dodici vittime, per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a lenire la sofferenza di quella comunità, sia mostrare lo spirito di condivisione nel merito rispetto alle proposte che dobbiamo alla comunità ischitana. Credo che, dopo la scorsa seduta nella quale abbiamo approvato importantissime risoluzioni che hanno visto un'Assemblea finalmente unita, anche in questa circostanza, al di là delle rispettive posizioni e sensibilità politiche, abbiamo la possibilità di dimostrare come l'Italia dinanzi al dolore si può far trovare coesa, solidale, finalmente unita. Questo lo dobbiamo alla comunità di Ischia, perché ha insegnato a ciascuno di noi cosa significhi il termine resilienza, e cioè la capacità di assorbire il colpo senza infrangersi e addirittura assorbire l'energia di quel colpo per affrontare le sfide del futuro. Questa ritrovata consapevolezza, che vede l'Aula sensibile al tema, deve arrendersi di fronte a un'evidenza che riguarda tutta la nostra Nazione, vale a dire che bellezza è anche fragilità e si è rotto quel rapporto che dobbiamo ricostruire tra natura e territorio, se è vero che il rapporto ISPRA parla del 97,9 per cento del territorio nazionale esposto al rischio di frane, alluvioni o di erosione costiera, e che addirittura circa il 20 per cento del territorio nazionale vede questo rischio elevato o molto elevato. Tuttavia, insieme all'orgoglio per il lavoro dell'Aula e per quello che è accaduto nell'altro ramo del Parlamento, dove questo decreto è stato convertito senza alcun voto contrario, per il lavoro nelle Commissioni per il quale ringrazio il senatore Fazzone e la senatrice Petrucci, sono profondamente orgoglioso anche di come ha lavorato e sta lavorando il Governo, che ha fornito in concreto un primo grande esempio di che cosa significhi buona politica, di che cosa significhi fornire risposte con un'immediatezza e un tempismo straordinari come si possa dare anche nel dramma una grande prova di efficienza e concretezza. La scansione dei tempi è stata significativa. Immediatamente dopo il dramma, già il giorno successivo c'è stata la decretazione dello stato di emergenza e, dopo cinque giorni,

il rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile. Ci sono poi stanziamenti molto importanti, per cui dai 17 milioni originari si è passati a oltre 85 milioni di contributi; una dotazione finanziaria di 40 milioni dal 2023 al 2026 di conto capitale per affrontare l'emergenza idrogeologica, mai prevista in passato. Oltre 20 milioni di fondi destinati alla rimozione dei fanghi, al loro smaltimento e alla loro caratterizzazione. Quel che conta, poi, per dimostrare il salto qualitativo nell'affrontare i problemi, è il rafforzamento con oltre 8 milioni della struttura di missione, con i conferimenti all'Autorità di bacino dell'Appennino meridionale. Questa è la cornice lungo la quale si sta muovendo il Governo: non più interventi episodici, non più misure

oltre che di mezzi, significa aver compreso che sulla dorsale appenninica meridionale c'è un unico tema che riguarda Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. *(Applausi)*. che il nostro ecosistema è talmente delicato da dover essere gestito con la debita attenzione è cristallizzato anche da due ulteriori elementi. elemento è che, quando si è trattato di individuare il Commissario straordinario, piuttosto che argomentare e abusare, come è stato fatto in passato, dello *spoils system*, si è deciso di attribuire i poteri commissariali allo stesso Commissario già incaricato di gestire il sisma del 2017, perché c'era la necessaria evidenza, al di là delle appartenenze politiche, di fornire in tempi brevissimi, con procedure snelle, i poteri commissariali al soggetto che in quel momento fosse il più idoneo ad affrontarli. La seconda circostanza è quella della struttura di missione, che in questo momento è l'unica possibilità che abbiamo di rafforzare il piano di assetto idrogeologico immaginato nell'ambito del decreto per stralci funzionali, che sono i più idonei a garantire la tutela del territorio. Non si tratta, quindi, soltanto di misure emergenziali, ma anche della prima prova di come va affrontato per il futuro, come finora non è stato fatto, il dramma della fragilità del nostro territorio. seguenti: aggiornamento degli strumenti di intervento e pianificazione; un nuovo metodo di lavoro - lo dico anche ai colleghi del MoVimento 5 Stelle - proprio alla luce dei criteri di previsione e prevenzione; revisione - come dicevano i colleghi di Forza Italia - del codice delle emergenze e del codice della procedura civile; soprattutto, immaginare un sistema preciso di attribuzione di responsabilità che per il futuro eviti il ricorso sistematico allo strumento commissariale. Bisogna, infine, definire un piano di protezione civile che coinvolga il territorio e sia quanto più possibile partecipato dalle comunità. Concludo, signor Presidente, immaginando che finalmente possiamo ritenere superato quel terribile aforisma di Prezzolini che diceva che in Italia non c'è nulla di più provvisorio del definitivo e nulla di più definitivo del provvisorio. Credo che, anche a partire dal decreto in esame, si possa comprendere come questo Governo stia costruendo una nuova Italia.

si possono evitare prima delle polemiche, prima di cercare i responsabili delle tragedie. Se si ha una struttura che serve a mettere in salvaguardia il nostro Paese, tutto quello che succede dopo alleggerisce anche le coscienze degli amministratori e dei politici che hanno fatto determinate scelte. Come diceva il poeta, la storia dà torto e dà ragione. il parere è contrario perché saranno adottati altri provvedimenti va anche contro quanto dichiarato, per esempio, dalla *premier* Meloni, che proprio su "Italia sicura" ha dimostrato un'apertura molto netta

mi spiace per chi si lamenta che qualcuno gli ha ricordato di averli cancellati. Ma la storia dà torto e dà ragione e chi ha cancellato questi strumenti ha delle grosse responsabilità anche oggi sul provvedimento esame, che magari non sarebbe stato così carico di dolore, ma avrebbe soltanto previsto dei risarcimenti in seguito all'avvenuta tragedia. esame non soltanto eroga dei soldi, ma soprattutto ci ricorda le vittime di quella circostanza che potevano essere evitate. Per

Fiumi di detriti sono scesi e hanno invaso il territorio, distruggendo case, macchine e strade, ma soprattutto progetti di vita e sogni di bambini. Ischia aveva bisogno di una risposta immediata e di strumenti per iniziare a guardare al futuro con speranza; così è stato. Tante le riflessioni: le mutate condizioni climatiche, il rapporto tra il territorio e i cittadini, la necessità di siglare un nuovo patto tra i diversi livelli di governo, di ammodernare la disciplina e la legislazione e di investire in tecnologia e innovazione, ma soprattutto in prevenzione e previsione dei rischi, in personale amministrativo e tecnico specializzato e qualificato. Alla fine sono stati destinati per l'isola 85 milioni di euro per interventi urgenti per le aziende, le famiglie e il territorio; cifra destinata nell'immediato a salire oltre i 100 milioni. Bisogna lavorare per cittadini informati, consapevoli fin dalla prima infanzia - come ha detto il capo del Dipartimento della protezione civile, l'ingegner Curcio - arrivare a un piano di protezione civile partecipato e vissuto da tutti, in fondo, per essere veramente attuato. Altro fattore sottolineato dallo stesso Curcio è la peculiarità idrogeologica dell'isola di Ischia e più in generale - aggiungo - le caratteristiche dei singoli territori italiani.

Non è pensabile sacrificare la nostra terra e, ancora peggio, i nostri cittadini a causa di una politica che volta le spalle alla responsabilità e alle scelte, talvolta impopolari, che devono essere compiute per il bene comune. È vero: dire di no non porta consenso elettorale, ma salva vite umane. Quella dell'urbanizzazione selvaggia è una piaga, se si pensa che il nostro Paese si costruisce erodendo suolo anche laddove il terreno presenta,

italiani (7.423 Comuni) è a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera. Ci vuole perciò prontezza di intervento in situazioni di emergenza dovute a calamità naturali, come garantito dal piano comunale di protezione civile che - secondo i dati del Dipartimento - sarebbe presente non in tutti gli 8.000 Comuni d'Italia, ma complessivamente in circa 7.000. È necessario lavorare affinché ogni Comune possegga e aggiorni il proprio piano emergenziale di protezione civile, perché questo deve essere pronto ad operare in caso di necessità e a salvare vite umane. È altresì necessario prevedere sistemi innovativi di allerta tempestivi e rapidi alla popolazione, come ad esempio un *sms* sul telefonino. Il Governo, nel disastro di Ischia, si è prontamente mosso, emanando un decreto per gli interventi in emergenza: non è rimasto a guardare, non ci ha pensato su, perché la vita delle persone deve venire prima di ogni altra logica politica. Ha quindi varato il provvedimento che a breve andremo a votare, sul quale tutta la nostra Commissione ha lavorato alacremente, un aiuto concreto alle popolazioni dell'isola di Ischia e un supporto per rialzarsi in vista della prossima stagione estiva, che porta con sé il turismo, settore fondamentale, anzi vitale, per l'economia di quest'isola meravigliosa. Certamente non si può pensare di avere tutto e subito, non in questi casi: sarebbe da irresponsabili. La soluzione ad un problema di questa portata deve prevedere un'azione pluriennale e strutturale ed è proprio in questa direzione che va il provvedimento del Governo.

cento dei Comuni italiani è a rischio di dissesto idrogeologico e, secondo l'ISPRA, sono 8 milioni gli italiani che vivono in aree ad alta pericolosità. Questi dati, così preoccupanti, indicano che ci troveremo certamente a gestire nuove emergenze. Questa non è un'ipotesi, ma una certezza, se il 94 per cento dei nostri Comuni è a rischio

per la prevenzione. Eppure in questi anni abbiamo deciso di affidarci all'economia dell'emergenza, perché forse è più proficua, e non all'economia della cura e della prevenzione.

di qual è il rischio idrogeologico su tutte le aree del territorio nazionale. Sono decenni che il Paese aspetta il completamento della cartografia geologica e, ancora una volta, gli unici Governi ad aver investito per riprendere il progetto di completamento della cartografia geologica sono stati i Governi Conte. *(Applausi)*. Abbiamo investito 25 milioni di euro, ma non sono sufficienti, perché ne servono

abbiamo provato a sollecitare tutte le altre forze politiche ad utilizzare parte dei fondi stanziati per la legge di bilancio per la cartografia geologica. Presidente, il risultato è stato che il MoVimento 5 Stelle ha utilizzato 6 milioni di euro dal proprio *budget*, che era affidato ai singoli Gruppi per la legge di bilancio, perché non abbiamo trovato nessuna altra forza politica

i nostri geologi, quelli che erano con noi in quest'Aula nella scorsa legislatura: il nostro compianto Franco Ortolani, il senatore Quarto, il senatore Coltorti *(Applausi)*, che per cinque anni, da geologi, si sono sgolati a dire quanto fosse necessario completare la cartografia geologica. Ma purtroppo questo strumento non è ancora a disposizione del Paese. Quali sono gli altri strumenti che possiamo utilizzare per la prevenzione? Intanto dobbiamo dotare i nostri Comuni di piani regolatori; gran parte dei Comuni italiani sono sprovvisti ancora oggi, nonostante tutte le tragedie, di piani regolatori. Dobbiamo contrastare l'abusivismo edilizio non solo con i proclami, ma con i fatti. Ricordo che anche su questo nella scorsa legislatura, nella delega fiscale, abbiamo fatto alla Camera un lavoro durato mesi. In quella delega fiscale c'era un primo passo verso il contrasto all'abusivismo edilizio: la digitalizzazione del catasto. Ma su questo punto il centrodestra ha alzato le barricate, accusando la maggioranza di voler mettere tasse sulla casa, quando non era assolutamente quello il punto. Il punto era:

emotivamente, in queste situazioni. Poiché non abbiamo fatto prevenzione e poiché non abbiamo utilizzato gli strumenti che avevamo a disposizione, ci siamo trovati ad affrontare un'ennesima tragedia, purtroppo annunciata. Il 26 novembre, alle 5 di mattina, dal monte Epomeo si è staccata una frana che ha inghiottito decine di case del Comune di Casamicciola e ha inghiottito e cancellato anche un piazzale dedicato ad Anna De Felice, la quindicenne che è morta a Ischia proprio in seguito a una frana nel 2009. Quindi dal 2009 nulla è cambiato e si è ripetuta esattamente la stessa tragedia, con numeri ancora più gravi, perché ci sono stati dodici morti La macchina per la gestione dell'emergenza si è messa subito in campo. Tutti i cittadini ischitani e campani e tutti i volontari si sono mobilitati, scavando a mani nude nel fango per giorni. I sindaci di Ischia hanno rivolto un appello al Governo a stanziare i fondi. Secondo la stima dei sindaci, servono 400 milioni di euro in un anno non solo per ripristinare lo stato delle cose, ma anche per mettere in sicurezza quel territorio. Invece noi oggi ci troviamo a discutere un decreto che stanzia appena un decimo di quelle risorse: solo 40 milioni di euro, tra l'altro spalmati in quattro anni, quindi 10 milioni all'anno, che - come dicono i sindaci, e noi condividiamo questa preoccupazione - non saranno sufficienti neppure per ripulire dal fango le strade e le case. E allora come sempre, Presidente, noi abbiamo provato a lavorare da opposizione in maniera costruttiva, proponendo degli emendamenti che avevano un unico scopo: scopo: alleggerire il carico per le imprese e per le famiglie del posto. Avevamo chiesto di cancellare imposte come la Tari, di sospendere le tasse universitarie e le rate dei mutui, di aiutare i Comuni permettendo l'assunzione di personale come sempre, questa maggioranza purtroppo dice di voler collaborare con le opposizioni, ma continua a dare solo pareri negativi e a bocciare tutte le nostre Evidentemente questa maggioranza spera solo nella resilienza della popolazione ischitana, che io sono convinta ci sarà anche questa volta. Quella popolazione, così come si è rialzata dopo la frana del 2009 e dopo il terremoto del 2017, si rialzerà anche dopo questa ennesima frana. Ma non possiamo continuare a dire ai cittadini che, tutto sommato, devono essere bravi a cavarsela da soli.

ci preoccupa la visione di questo Governo sul contrasto al dissesto idrogeologico. Ci preoccupa perché in legge di bilancio, Presidente, sono state tagliate il 40 per cento delle risorse che erano destinate al dissesto idrogeologico. Ci preoccupa perché questo Governo ha deciso di riprendere a trivellare i nostri fondali e sappiamo quanto questo sia pericoloso proprio per il dissesto idrogeologico. Ci preoccupa perché dal programma di questo Governo è stata totalmente cancellata la transizione ecologica, che era invece uno dei pilastri su cui abbiamo costruito il PNRR. Quindi, è chiaro che per questo Governo e per questa maggioranza l'emergenza climatica non è reale; è chiaro che il contrasto ai cambiamenti climatici non è l'emergenza più importante che deve gestire questo Paese. Quello che non è chiaro a questa maggioranza e a questo Governo è che veramente non c'è più tempo per invertire la rotta. Bisogna dire basta all'utilizzo dei combustibili fossili e anche basta a tutti quei sussidi ambientalmente dannosi, i cosiddetti SAD, per i quali spendiamo ogni anno 21 miliardi di euro. Noi, Presidente, spendiamo 21 miliardi di euro praticamente per foraggiare, pagare e incentivare la nostra stessa estinzione. Questo è quello che stiamo facendo, quando invece quelle risorse andrebbero utilizzate tutte per una transizione ecologica vera, per investire nelle rinnovabili e per mettere davvero in sicurezza questo nostro fragilissimo Paese.

Ovviamente non siamo insensibili ad alcuni punti che pure sono contenuti nel decreto-legge, ma non possiamo non sottolineare come questi rappresentino

perché le cifre stanziate che sono spalmate negli anni - come sappiamo - sono largamente inferiori a quello che occorrerebbe, ma soprattutto perché il il provvedimento sembra, ancora una volta, ispirato ad una logica puramente emergenziale, senza alcun tentativo, cioè, di cominciare a dare qualche risposta strutturale che servirebbe evidentemente non soltanto all'isola di Ischia, ma più in generale per ragionare su una tendenza da perseguire nell'intero Paese. Le risorse stanziate, 40 milioni di euro, sono insufficienti. Sappiamo che le richieste fatte dall'isola di Ischia - com'è stato ricordato adesso - per il solo primo anno, per interventi di messa in sicurezza del territorio e di riqualificazione ambientale, parlano di circa 400 milioni di euro, cifre assai lontane da quelle previste. Sono state anche ricordate le audizioni che ci sono state in Commissione dei sindaci e le loro richieste disattese. Naturalmente auspico che quello di oggi sia soltanto un primo passo, ma purtroppo devo dire che ho dei dubbi. Temo che non sarà così, anche perché l'isola di Ischia - come sappiamo - è stata soggetta, negli ultimi vent'anni, ad una serie di tragedie dovute ad eventi temporaleschi tipicamente tropicali, fenomeni che fino a pochi anni fa non erano parte del sistema climatico del nostro Paese. Si tratta di eventi che sono intervenuti - com'è noto - in un territorio particolarmente fragile, devastato dagli abusi e dall'incuria. Vorrei ricordarlo: peraltro parliamo di un'isola che ha

avrebbe potuto rappresentare davvero in maniera diversa rispetto al passato un modo finalmente nuovo di affrontare la questione di cui stiamo discutendo, evitando cioè di cadere nella solita ed esclusiva lettura emergenziale e provando invece ad immaginare una qualche risposta strutturale. Invece, come sempre, rincorriamo le emergenze, dimostrando ancora una volta di non voler affrontare la realtà per quella che è, peraltro dimenticando che la tragedia che ha colpito l'isola di Ischia è l'ennesimo frutto avvelenato davvero di un combinato disposto: da una parte il cambiamento climatico, dall'altra l'incuria del territorio. cambiamento climatico aumenta a dismisura i fenomeni estremi, come si vede anche in queste ore e come si è visto in tutti questi mesi, alternando una siccità straordinaria a fenomeni meteorologici estremi. Si tratta però - badate bene - di un cambiamento climatico che in tutto il mondo le destre - che in questo Paese governano l'Italia - hanno totalmente negato nel corso degli anni; hanno minimizzato,

vi indignate, come abbiamo visto, in maniera molto forte per la vernice lavabile e avete invocato anni e anni di carcere per gesti che possono essere più o meno sbagliati, ma che comunque restano dimostrativi e non violenti, però poi non battete ciglio, anzi voltate la faccia completamente dall'altra parte, rispetto a quegli studi scientifici

dall'inizio dell'anno ci sono stati diciotto eventi climatici estremi e sono ben cento quelli monitorati dal 2010 al 2020; ci sono state trentotto alluvioni e quattro frane: tutti fenomeni purtroppo nuovi, eventi estremi che provocano ovviamente morte e danni economici molto ingenti. L'Agenzia europea per l'ambiente stima una cifra in trent'anni pari a 75 miliardi di danni soltanto per il nostro Paese, mentre naturalmente in termini di vite umane questo bilancio è ancora più drammatico, poiché ci parla di 279 vittime nell'ultimo decennio e 29 nello scorso anno (più di quelle precedenti). Insomma, è un bollettino davvero devastante,

di combinato disposto perché, assieme al cambiamento climatico, l'altra grande questione che va nominata si chiama incuria del territorio. Questo non solo a causa dell'assenza di prevenzione, che pure ci consentirebbe di risparmiare l'80 per cento delle cifre che di volta in volta stanziamo, esattamente come stiamo facendo adesso (al di là del fatto che queste risorse siano sufficienti o meno), ma anche perché, purtroppo ancora una volta, alcuna centralità a quegli interventi legislativi che invece occorrerebbe mettere al centro dell'iniziativa politica: la legge sul consumo di suolo, per citare la prima iniziativa che ci viene in mente e che aspettiamo invano da due legislature; la legge per il clima, cioè uno strumento normativo in grado di fissare finalmente degli obiettivi vincolati. Non si tratta solo dell'assenza di un intervento strategico, capace di prevenire e non soltanto di tamponare, per così dire, l'emergenza, ma anche dell'incuria del territorio che - diciamocelo nella maniera più chiara possibile - è stata la cifra ricorrente di anni e anni di politiche scellerate, esattamente come quei condoni edilizi e quelle sanatorie di edifici realizzati spesso nelle aree a rischio idrogeologico, condoni che però non sono stati fatti senza che ci fosse un ritorno, ma su cui invece sono stati costruiti veri e propri sistemi di potere, filiere di preferenze. L'ho già detto alcune settimane fa, durante l'informativa resa dal Ministro immediatamente dopo la tragedia e lo ripeto ancora una volta oggi: pochi mesi fa in Campania, durante la campagna elettorale, alcuni partiti oggi

pochi decenni fa e guarda caso sono gli stessi partiti che minimizzano oppure negano in radice il cambiamento climatico. Si continua a perseguire questa linea, pensando di costruire politiche energetiche ancora basate sulle fonti fossili, si fanno le crociate contro le case *green*, si vuole trivellare il mare e anche nel provvedimento in esame - come dimostrano gli stessi emendamenti che abbiamo presentato e che sono stati respinti, prima alla Camera e oggi qui in Senato - si vede chiaramente come si continua a strizzare l'occhio, fatemi dire così, a quelle forme di abusivismo che evidentemente ancora rappresentano un serbatoio di voti. Se, per esempio, le ordinanze di demolizione non vengono eseguite nelle zone rosse, rosse, già solo questo dato imporrebbe in un decreto come questo di immaginare interventi capaci di evitare il ripetersi di queste situazioni; sono stati invece respinti per l'appunto quegli emendamenti in cui si chiedeva di dare alle prefetture la possibilità di ottemperare

Per tutte queste ragioni, che attengono all'efficienza degli strumenti proposti, da una parte, ma più in generale anche al taglio del provvedimento, non voteremo a favore del disegno di

rappresentante del Governo, colleghi, intervenire *ex post* nelle situazioni di dissesto idrogeologico, quando ci sono stati consistenti danni alla popolazione e morti, è doveroso e quindi il Gruppo per le Autonomie sosterrà questo provvedimento. di aggiungere qualche riflessione. Innanzitutto, tra un paio di settimane in quest'Aula esamineremo un provvedimento simile, che riguarderà le alluvioni nelle Marche, il terremoto di L'Aquila, provvedimenti conseguenti ad altri disastri ambientali. Siamo sicuri che sia efficiente ed efficace a così stretto giro avere più provvedimenti che arrivano all'esame di quest'Aula? Io non credo, ma evidentemente la maggioranza ritiene che sia così. Viviamo in una crisi climatica drammatica - ed è una crisi, non si può parlare solo di cambiamenti, cari colleghi ed è quindi evidente che bisogna assumere provvedimenti di prevenzione, il che significa vincolare beni immobili spesso privati. Tuttavia, in un Paese ad altissima concentrazione di avvocati come l'Italia è difficilissimo che si riesca a porre questi vincoli in tempi ragionevoli, perché, come è giusto che sia, il proprietario che si vede limitato nella possibilità di godere andrà in tribunale, con tempi e costi che spesso le amministrazioni locali non sono in grado di sostenere. Una riflessione su questi aspetti, quindi, va fatta. Non possiamo poi prendercela con i sindaci perché non sono stati in grado. Sono non sono stati in grado. Sono stati fatti anche i condoni, ma gli edifici realizzati abusivamente per essere abbattuti necessitano di provvedimenti che possono essere impugnati. Qui si tratta di dare un taglio abbastanza chiaro dal punto di vista normativo a questo tipo di situazioni. Non vedo movimenti nell'area del Governo che portino verso questa direzione e credo che sia invece assolutamente necessario prendere in mano in questo senso la situazione. Il senatore De Cristofaro, che mi ha preceduto, ha ritenuto di addossare la responsabilità a una certa facilità con cui la destra nel mondo non affronta questa tematica. Credo, però, che il nostro sia un Paese che ha una ragionevolezza di fondo e quindi mi auguro L'Italia è notoriamente il Paese dell'improvvisazione, siamo famosi perché nelle difficoltà sappiamo tirar fuori il meglio di noi stessi. che a qualche forza politica venisse in mente di non fare nulla o di fare poco perché paga di più avere gli eroi che intervengono dove ci sono stati i disastri che non vincolare, come detto prima, beni immobili dei cittadini che in tal modo si trovano a non essere favorevoli a quella forza politica che ha preso quel provvedimento. Queste sono le riflessioni che volevo fare, ma ribadisco che il Gruppo per le Autonomie voterà a favore di questa norma. nostro esame arriva blindato al Senato, che non l'ha potuto analizzare in maniera compiuta apportando le migliorie che tutti i Gruppi parlamentari avrebbero voluto realizzare.

pochi ma subito - alcuni finanziamenti per l'emergenza. Noi li avremmo voluti in conto corrente, cioè come spesa immediata, e non in conto capitale, capisco che è arrivato in un momento di passaggio, con la legge di bilancio, e quindi probabilmente le risorse non c'erano. L'emergenza, però, rischia di prolungarsi anche dal punto di vista del recupero del territorio. appunto il decreto riguarda solo la parte emergenziale e non si percepisce nulla su interventi di carattere strutturale. Mi ha preceduto un collega che è stato sindaco e quindi sa cosa vuol dire per i sindaci avere degli strumenti adeguati per realizzare quella tutela del patrimonio naturale che spesso i piccoli Comuni non hanno. Questo è un Paese che continua a spendere tantissimo nell'emergenza e pochissimo nella prevenzione e quando ha degli strumenti per la prevenzione del MoVimento 5 Stelle che in discussione generale ha accusato il senatore Renzi di aver gettato fango sul MoVimento, vorrei ricordare semplicemente le parole del Presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, non proprio ascrivibile al *club* renziano, che ha denunciato come l'articolo 25 del cosiddetto decreto Genova fosse un condono vergognoso su Ischia.

non si può pensare che i piccoli Comuni mettano in salvaguardia il patrimonio naturale con i geometri dei Comuni. L'unità di missione "Italia sicura"serviva a fare una cabina di regia nazionale per far spendere i soldi locali attraverso l'azione delle Regioni e degli enti locali. Per questo, signor Sottosegretario, mi è dispiaciuta la sua la sua contrarietà all'ordine del giorno, che noi riproporremo come emendamento al nuovo decreto, facendo di questa la nostra battaglia. Piangere le vittime dopo, infatti, è alquanto ipocrita, se non si

bisogna sdoganare un provvedimento che non vede mai la luce. Questa, in maniera assolutamente fortuita, è la mia terza legislatura. Eppure, è dal 2013 che vedo arenarsi la legge sul consumo del suolo. un fenomeno che non può più accadere in questo Paese. Noi continuiamo a consumare suolo agricolo per costruire come se fossimo in un *boom* economico e di popolazione. Purtroppo, il nostro Paese non è più in una situazione di crescita natale che giustifichi una continua costruzione da terreni vergini. allora mettere un argine definitivo, sia per ciò che riguarda l'abusivismo, ma soprattutto per quanto riguarda la costruzione dal nuovo in questo Paese. Grazie ai criteri che ormai la scienza ci non è più casuale non costruire in alcuni luoghi. Abbiamo ormai tutte le conoscenze per sapere che, se si costruisce in zone esondabili, sicuramente si va incontro a problematicità incredibili; che, se si costruisce in terreni fragili, si rischia la vita di chi abita in quei luoghi. I futuri decreti, che noi vogliamo non solo per Ischia ma per l'intero nostro patrimonio e per la salvaguardia territoriale, devono prevedere degli strumenti adeguati per mettere in sicurezza il nostro patrimonio edilizio, per mettere in sicurezza i nostri fiumi, per mettere in sicurezza le nostre terre, ma soprattutto per smetterla di continuare a costruire in modo indiscriminato. Noi abbiamo intere aree ormai in disuso industriale. Dobbiamo fare delle politiche fiscali perché il recupero di quelle aree convenga molto di più che non costruire sul nuovo. Se il Governo farà queste misure, noi come Azione-Italia Viva-RenewEurope saremo dalla vostra parte, perché la nostra è un'opposizione dura, quando non fate le cose; quando, invece farete delle cose per il Paese, noi saremo al vostro fianco, con idee e con proposte, come quella di far ritornare l'unità di missione "Italia sicura". Essa ha funzionato: lo dicono i fatti, lo dicono i luoghi, lo dicono le strutture che sono state realizzate.

Per dare una risposta a quei territori che in questo momento stanno guardando al Parlamento con grande ansia e preoccupazione, non daremo un voto contrario. Ci aspettiamo qualcosa di meglio nei prossimi decreti

la conversione in legge del decreto-legge recante interventi relativi ai danni provocati dalla catastrofe alluvionale dello scorso 26 novembre. Ancora una volta questo Governo ha mostrato velocità e determinazione nell'affrontare il dramma di una calamità naturale che ha colpito una delle più belle isole d'Italia; una soluzione ai problemi voluta nell'immediato dall'Esecutivo e migliorata dal lavoro della Camera, che ha esaminato il provvedimento in prima lettura. Siamo riusciti in tempi *record* a stanziare circa 85 milioni di euro per i primi necessari interventi per la popolazione dei Comuni colpiti da quella brutta emergenza. L'ambito degli interventi del decreto-legge è stato, infatti, ampliato dopo le informazioni raccolte durante l'esame da parte della Camera e dopo una lunga serie di audizioni in cui si è entrati nel merito dei problemi e delle soluzioni. In effetti, diversi In effetti, diversi sono gli articoli aggiunti al testo iniziale del decreto-legge, che tengono conto delle soluzioni proposte; un testo che, oltre al numero di articoli e alle previsioni degli interventi, ha visto crescere anche i fondi a disposizione, fino ad arrivare a 85 milioni di euro.

abbia fatto e stia ancora facendo per la nostra isola, con l'obiettivo di garantire un intervento concreto, e non solo per la recente alluvione, ma anche per i danni causati che ha colpito la città di Casamicciola nel 2017. Si consideri che Ischia in tutta la sua storia ha subito ben 13 eventi sismici. Insomma, per tutti questi anni gli amministratori e i cittadini di Ischia hanno dovuto subire i tanti *slogan* di una politica che poco ha compreso le problematiche di quel territorio, ma soprattutto che nulla ha prodotto in termini di sostegno per un'isola che dovrebbe essere un fiore all'occhiello per il settore turistico del nostro Paese. Gli interventi che sono stati messi in campo e previsti negli 85 milioni di euro vanno nell'esclusivo interesse del territorio e dei cittadini che vivono in quelle zone. La *ratio* del decreto-legge e delle sue successive modifiche è stata proprio quella di coinvolgere tutti gli attori interessati. Per questo si sono recepite le proposte e le istanze di tutti coloro che hanno saputo e potuto apportare un contributo concreto: la struttura commissariale, l'Autorità di bacino, gli amministratori locali, i tecnici e tutti coloro che partecipano a vario titolo alla ricostruzione, ma anche coloro che sono stati individuati per ridare subito operatività al tessuto economico e sociale dell'isola. Questo è stato il senso della iniziale sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, ma anche del rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali e la parallela sospensione delle udienze e dei termini processuali per i giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari. Saranno reclutate nuove unità per rafforzare l'Autorità di bacino; sarà rifinanziato il fondo regionale della prevenzione civile; partirà il piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione e ci saranno tante altre misure urgenti in favore della popolazione e dei Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi alluvionali e franosità Grazie a tutti Forza Italia non può che essere soddisfatta delle misure previste nel decreto-legge, necessario e fin troppo urgente per una popolazione che per troppo tempo è rimasta nel dimenticatoio e che ha visto nel periodo *post* terremoto, nel decreto-legge cosiddetto Genova, l'unico intervento dello stesso Governo Conte, Conte, in cui veniva prevista una sanatoria per la ricostruzione di Ischia, senza entrare nel merito delle problematiche inerenti a un territorio così complesso e geologicamente unico. Per questo motivo non possiamo che essere soddisfatti del lavoro puntuale e preciso di questo Governo e Ischia può davvero sperare finalmente in una nuova stagione. Eravamo certi della ripresa dei tanti cittadini dell'isola. Ma, se vogliamo che il Paese si rialzi, è necessario programmare e stanziare fondi conoscendo le problematiche che si vanno ad affrontare. Non sono servite passerelle e non serviranno proclami. Ischia è nel cuore di questo Governo e di Forza Italia, che lavorano quotidianamente e lontano dai riflettori. Quello che ci sta a cuore è soprattutto mettere gli amministratori locali nelle condizioni di operare al meglio, potendo contare sulle risorse dello Stato. Noi crediamo che le misure di questo decreto-legge potranno iniziare a restituire agli ischitani la certezza di tornare a condizioni di vita normale e soprattutto a competere con la loro straordinaria accoglienza sul versante dell'offerta turistica mondiale. Saremo ancora dalla loro parte e, come Gruppo Forza Italia, votiamo convintamente a favore del provvedimento. Signor Presidente, gentile Sottosegretario, colleghi, parlando oggi del provvedimento che riguarda le popolazioni di Ischia, credo che due premesse siano d'obbligo.

Ischia rappresenta, con oltre 4 milioni di presenze nel 2019, ultimo anno di turismo forte in Italia, il punto più importante per la Campania per quel che riguarda il PIL nel settore turistico. La seconda premessa è una provocazione.

il cambiamento climatico o l'abusivismo edilizio, che sono dei problemi che esistono, ma che purtroppo nulla hanno a che vedere con la tragedia che ha colpito l'isola di Ischia. Ho già detto in quest'Aula e in altre sedi che altre alluvioni che hanno caratterizzato quest'isola purtroppo sono avvenute nel 1557, nel 1662, nel 1762, nel 1767, nel 1796, nel 1827, nel 1841 e nel 1863. Tutto questo dimostra che i temi e le strumentalizzazioni ideologiche servono a poco perché la popolazione ischitana e gli amministratori sono le vittime e non i colpevoli di questa tragedia; tragedia che - a detta dei geologi che abbiamo sentito - sarebbe stata evitabile solo se ci fosse stato un muro largo 28 metri; immaginate un muro di 28 metri per fermare la massa scesa dal monte Epomeo verso valle.

della necessità di pianificare. La Regione Campania ha 339 milioni di euro a disposizione

della necessità di pianificare. Ricordo, prima di tutto a me stesso, che nel 2017 c'è stato un sisma ad Ischia. La prima Conferenza dei servizi c'è stata il 24 ottobre del 2022. Cinque anni dopo il

Con quei tre milioni non sono stati predisposti neanche progetti. Su quattro miliardi di fondo sociale europeo, a disposizione della Regione Campania da nove anni, ne abbiamo utilizzati meno della metà. E allora non diamo le responsabilità ai cittadini e agli amministratori. Nel 2018 il segretario della Lega Matteo Salvini mi chiese di accompagnarlo sull'isola per vedere i disastri prodotti dal terremoto. E ci siamo recati nuovamente a inizio gennaio per renderci conto in

con il primo Consiglio dei ministri a settantadue ore dal 26 novembre, proclamando lo stato di emergenza, nominando un commissario, stanziando i primi fondi e sospendendo i tributi. Vengo a questo decreto-legge, che richiede due premesse. In merito alla prima, un ringraziamento va alle minoranze, e uso volutamente il termine minoranze e non opposizione, perché - come mi è stato detto dai miei colleghi del Gruppo Lega della Camera - hanno collaborato in Commissione alla Camera per arrivare a una soluzione quanto più condivisa.

che c'è bisogno di piani di prevenzione del rischio idrogeologico quando sono a disposizione 339 milioni da nove anni. Ci sono 339 milioni a disposizione e ne è stato speso solo il 20

- il rischio di idrogeologico riguarda e accomuna tutta l'Italia meridionale - e, come se non bastasse, è passato un ordine del giorno alla Camera, a firma di tutto il centrodestra unito, che chiede un impegno al Governo, che ha dato parere favorevole, a uno stanziamento di ulteriori 25 milioni. È tutto ciò che serve? Assolutamente no, ma abbiamo fatto quello che potevamo fare, considerando il periodo, il conflitto russo-ucraino e lo stato di emergenza. Si tratta di una pronta e iniziale risposta che è stata percepita dagli ischitani in maniera più che positiva, e noi come Lega torneremo sull'isola di Ischia già la settimana prossima per ascoltare le loro risposte. Un'altra misura importante è stata la proroga della chiusura della sede distaccata del tribunale di Ischia di Ischia per un altro anno. Questo è un problema che riguarda non solo l'isola di Ischia, ma anche l'isola d'Elba e l'isola di Lipari. E mi auguro che, quando si parlerà di riforma della geografia giudiziaria, i tribunali isolani trovino una una stabilizzazione perché sono dei punti di legalità in queste isole. Quindi, auspico una soluzione definitiva e non più tampone. Da ultimo, una richiesta che proveniva dall'isola di Ischia - e l'abbiamo recepita nel decreto-legge - era uniformare le procedure previste dal commissariamento del terremoto del del 2017 e quelle previste dal commissariamento per l'alluvione del 2022. È assurdo che, per una stessa strada interessata dal terremoto e dall'alluvione, fossero previste due procedure diverse, per cui siamo diventati l'ufficio complicazioni delle cose semplici; cose semplici; questo semplicemente per una presunzione di colpevolezza perenne, da parte degli amici del centrosinistra, contro gli imprenditori, contro gli amministratori locali. allora che, invece di essere l'ufficio complicazioni delle cose semplici, questo Parlamento, l'attuale Governo e la sua maggioranza diventino l'ufficio semplificazione delle cose complicate. Per questo annuncio il voto favorevole della Lega. Signor Presidente, gentile Sottosegretaria, senatrici, senatori, non c'è spazio, di fronte a quello che è accaduto il 26 novembre scorso a Ischia, per la polemica politica vuota e pregiudiziale. Abbandonarsi ad essa sarebbe una cinica mancanza di rispetto verso le dodici vittime, tra le quali un bambino di soli ventidue verso i feriti, gli sfollati, ma anche verso coloro ai quali abbiamo rivolto parole di gratitudine da questi banchi, con la senatrice Valente, il 1° dicembre. Ribadiamo ancora la più profonda gratitudine verso i soccorritori, i volontari, gli angeli del fango, le Forze di polizia, i Vigili del fuoco, i medici, i tecnici e tutta la comunità civile e istituzionale che ha reagito con orgoglio e forza all'ennesima tragedia. perché in soli tredici anni i cittadini di Casamicciola hanno affrontato due alluvioni e un terremoto, a cui si aggiungono ovviamente il collasso pandemico e la crisi economica. Dobbiamo a tutti loro, quindi, uno spirito collaborativo, privo di partigianeria, che condivida le finalità scritte nel provvedimento in esame. Per questo ci asterremo, ma

li avete respinti, perché di fatto ci siamo acconciati a una specie di "doppio monocameralismo". Per ragioni di tempo, si approva quello che è stato già discusso nell'altro ramo del Parlamento. Accogliamo quindi l'apertura, da parte della maggioranza, a valutare il merito delle nostre proposte, nella discussione che si è avviata per la conversione del decreto-legge interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, come d'altra parte ha detto il presidente Fazzone. Avrebbe forse avuto senso, come ha detto il senatore Spagnolli, fare un unico provvedimento, ma così è. Per noi non è importante di che colore sia la legge, l'importante è che "prenda" - diciamo così - la soluzione dei problemi. Onorevoli colleghi, sapete che i problemi che abbiamo indicato sono reali, intanto perché emergono dal territorio da chi li vive sulla propria pelle, a partire dagli amministratori locali, che sono in gran parte di centrodestra: parlateci! Poi abbiamo ascoltato i commissari: la commissaria prefettizia Simonetta Calcaterra e il commissario Giovanni Legnini. A tal proposito, si pone un tema di metodo, come ha giustamente detto proprio ieri il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, audito in 8a Commissione. Egli ha detto che il Governo si deve fidare dei commissari che esso stesso nomina o delle proprie articolazioni locali. È vero, non possono essere una controparte. Ebbene, tutti questi soggetti dicono innanzitutto che le risorse sono largamente insufficienti. Il "decretino" varato dal Governo, prima di arrivare in Parlamento, stanziava 17 milioni di euro. Oggi abbiamo una "leggina",

Prendo in prestito una formula che in quest'Aula usò il senatore Carlo Levi, rivolgendosi, nel 1969, al Governo Rumor, un Governo monocolore, come pian piano tende a diventare anche quello in cui un partito oscura vieppiù gli altri. È anche un Governo diminutivo, perché i fatti tendono a essere sempre in sedicesimi rispetto alle promesse, quando non a marcia indietro o in contraddizione, come ha detto bene il senatore Irto, proprio in relazione a quanto stiamo discutendo sul codice degli appalti. In questo caso, che le risorse siano insufficienti lo sapete anche voi, onorevoli colleghi. Quando alla Camera dei deputati si è discusso l'ordine del giorno dell'onorevole De Luca, che impegnava il Governo a trovare più risorse, il Governo ha dapprima reagito chiedendo di trasformare l'ordine del giorno in semplice raccomandazione. Nel dibattito si è poi ravveduto. Anche qui abbiamo approvato infatti più risorse, proprio per fare quello che abbiamo proposto: affrontare con urgenza la sistemazione temporanea delle famiglie e prevedere un contributo per chi le ospita. Ancora cinque giorni fa l'allerta meteo arancione ha comportato un'ulteriore evacuazione: oltre a coloro che vivono nelle zone a rischio di Casamicciola, sono state allontanate anche 90 persone dalla zona di Monte Vezzi, ad Ischia Porto, altra località su cui grava il rischio idrogeologico e dove nel 2006 si verificò una frana, nella quale persero la vita altre quattro persone. impegnare 3 milioni e non 1,7, per assicurare al Comune il gettito dei tributi non versati, altrimenti - uso le parole della commissaria - il Comune sarà impossibilitato a offrire i servizi essenziali. intervenire per i mancati introiti della Tari e sospendere l'Imu sulle abitazioni inagibili, com'è stato fatto per altre calamità, sospendere i mutui MEF e rifinanziare il fondo della protezione civile, non con 10, ma con almeno 50 milioni di euro, stanziare almeno mezzo milione per il trasporto scolastico e prevedere un ristoro per le aziende agricole e le altre attività economiche. Occorre riflettere sull'istituzione di una zona franca urbana, coprire il buco di bilancio dei Comuni, com'è già stato fatto per L'Aquila, per l'Emilia e per il centro Italia, colpiti dai rispettivi terremoti, e soprattutto aiutare chi era prima degli eventi, perché forse non esisteranno più le classi sociali, ma le calamità restano di classe e colpiscono sempre con maggior durezza i più poveri.

lo sviluppo sostenibile (CIPESS); solo alla Campania spettano 5,6 miliardi, usiamo quelli. E soprattutto facciamo quello che già abbiamo discusso e condiviso, almeno come intento, in Commissione: lavoriamo a un codice della ricostruzione che stabilisca un metodo di intervento applicabile sempre evitando di far sentire alcuni territori - o, se preferite, alcune tragedie - di serie B. Re-istituiamo presto l'unità di missione "Italia sicura", così come previsto dall'ordine del giorno approvato qui il 14 dicembre; prima ancora, coniughiamo la risposta a un'emergenza con una strategia che prevenga i problemi, invece che inseguirli. Che altro deve accadere per renderci tutti consapevoli che siamo su un piano inclinato? Davvero - come avrebbe detto Gramsci - la storia insegna, ma non ha scolari? stato già detto alla Camera, l'Agenzia europea dell'ambiente ha calcolato nel nostro Paese 1.503 eventi climatici estremi negli ultimi dodici anni, 780 Comuni colpiti e 279 vittime; ma di attenzione, 310 eventi e 29 morti ci sono stati solo nel 2022. Stiamo parlando di 75 miliardi di euro di danni negli ultimi quarant'anni (l'ha già detto il senatore De Cristofaro). Capite bene che, paradossalmente, le risorse per Ischia, che sono poche, sarebbero persino inutilmente troppe se si potesse prevenire, con una strategia più netta di adattamento e mitigazione del caos climatico, accelerando la transizione ecologica dell'economia. Voglio ringraziare tutte le senatrici e i senatori, ma anche le deputate e i deputati di maggioranza e di opposizione, che hanno condiviso la proposta di istituire una Commissione d'inchiesta bicamerale sugli effetti dei cambiamenti climatici, per essere tutti più consapevoli e capaci poi di dare forma a scelte politiche più chiare e non ideologiche, come ad esempio serve per quanto riguarda il Piano nazionale di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. L'altro elemento è la buona gestione del territorio. Nel nostro Paese manca ancora una legge contro il consumo del suolo. Da quando è iniziata la discussione questa mattina, alle 10,07 circa, sono stati consumati in Italia quasi 20.000 metri quadri di suolo, 2,2 metri quadri al secondo. Per questo l'ISPRA ci dice dati del 2021, oltre 540.000 famiglie e 1,3 milioni di abitanti vivono in zone a rischio frane, mentre ci sono 3 milioni di famiglie e quasi 7 milioni di abitanti residenti in aree a rischio idrogeologico. Siamo arrivati a una media di quasi 3 miliardi l'anno di danni per frane e alluvioni,

La strada opposta a tutto questo qual è? È quella dell'abusivismo e dei condoni. Già in quest'Aula abbiamo ricordato chi li ha promossi e chi li ha approvati; essi sono il miglior modo di scavare un pozzo senza fondo di disastri, dolore e risorse necessarie a "emergenze strutturali", se si può usare questo ossimoro. Allora conviene davvero «tenere altro viaggio», «ché questa bestia» - richiamando una famosa terzina del primo Canto - «ha natura sì malvagia e ria, / che mai non empie la bramosa voglia, / e dopo 'l pasto ha più fame che pria» (così abbiamo anche reso omaggio a un illustre padre della destra italiana).

che non è chiamato a essere un nobile commentatore di quello che viene deciso alla Camera. Lavoriamo su quello che manca, aiutiamo il Governo diminutivo a essere non dico superlativo, ma giusto, coerente e lungimirante. *(Applausi)*.

Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, intervengo in rappresentanza del Gruppo Fratelli d'Italia e da campano sono onorato di poterlo fare su un provvedimento così importante come il decreto Ischia. Le immagini della frana hanno agghiacciato il cuore di ognuno di noi e consentitemi di esprimere, anche da quest'Aula, la mia e la nostra solidarietà e vicinanza ai cittadini residenti ad Ischia. Da subito, il presidente Meloni e il Governo hanno rivolto sentimenti di gratitudine ai soccorritori, a quei giovani che non si sono risparmiati per aiutare le vittime di quell'eccezionale alluvione: dalla Protezione civile ai suoi volontari, dai Vigili del fuoco agli operatori intervenuti per prestare assistenza e supporto alla popolazione, ci hanno fatto sentire tutti una comunità ancora più orgogliosa di far parte della grande famiglia Italia. Grazie a tutti per lo sforzo immane messo in campo nelle ore successive al disastro, che ancora sta continuando. un disastro idrogeologico che fa male a tutta la Nazione, perché l'isola di Ischia, con le sue bellezze naturali, rappresenta un patrimonio inestimabile, direi un patrimonio dell'umanità, che contribuisce a rendere grande il nome dell'Italia nel mondo. Proprio su un tema così delicato, che ha causato tanta disperazione e tanta sofferenza, non possiamo accettare alcune strumentalizzazioni e sterili contrapposizioni che arrivano da una parte dei dirimpettai; certo, servono più prevenzione e meno emergenza, ma chi ha avuto più tempo per programmare azioni di prevenzione oggi lamenta la mancanza delle azioni in tal senso. Qualcosa non va per il suo verso. Se dovessi inseguirvi sulla strada della polemica, oggi dovrei sottolineare qualche provvedimento del passato, ma mi asterrò dal farlo, perché mi battereste sull'esperienza. Piuttosto che la polemica, invece, i cittadini di Ischia si aspettano delle risposte e noi le abbiamo date e continueremo a darle. Oggi, quindi, vogliamo tutti ringraziare il Governo Meloni per la concretezza dimostrata e per porre l'accento sulle azioni che questo Esecutivo ha messo in campo e si accinge ancora a fare. La maggioranza ha assunto degli impegni e, con coerenza, sta lavorando per onorarli. I Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali e franosi che, a partire dal 26 novembre, hanno causato vittime e determinato una grave situazione di pericolo, con il conseguente isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, hanno ricevuto immediato sostegno già nelle prime ore di emergenza. La stessa sera del 26 novembre, nell'immediatezza degli eventi, sono stati stanziati 2 milioni di euro per le esigenze primarie. Il Governo, di fronte a una catastrofe naturale così importante, ha agito rapidamente, rispondendo alle necessità e ai bisogni urgenti delle popolazioni colpite. Dopo soli cinque giorni, il Consiglio dei ministri, con un secondo intervento, ha disposto l'erogazione di altri fondi oggi finalmente, con la conversione in legge del decreto-legge n. 186, aumentiamo ancora le risorse da destinare all'isola, prevedendo uno stanziamento non di 40 milioni di euro (quello riguarda solo una parte dei fondi messi a disposizione nel piano 2023-2026), ma di oltre 85 milioni di euro, ai quali andranno sommati, nell'immediato futuro, altri 25 milioni che il Governo, approvando un ordine del giorno, si è impegnato a reperire per fronteggiare l'emergenza. Sappiamo che la situazione resta delicata e va continuamente monitorata, ma terremo alta l'attenzione e, qualora tali risorse non dovessero bastare, saremo pronti a intervenire nuovamente e in modo più incisivo. Condividiamo le parole del ministro Musumeci: per Ischia e per altri territori a rischio c'è bisogno di uno studio approfondito, volto ad affrontare il problema su scala nazionale, attraverso interventi strutturali a tutela dell'ambiente per preservare i nostri territori e proteggere i cittadini. Siamo al lavoro per tutelare e sostenere anche il comparto economico dell'isola. Intendiamo mettere in campo azioni concrete, che siano da spinta per il rilancio del settore turistico e culturale. Nella stessa direzione le parole del ministro Garnero Santanchè sull'impegno del Governo a una campagna di promozione straordinaria per esaltare i tratti caratteristici dell'isola e le sue bellezze naturali. Dopo il cordoglio per le vittime dell'alluvione, il Governo, l'intero consesso parlamentare e noi di Fratelli d'Italia abbiamo affrontato e stiamo affrontando il problema con competenza, pragmatismo e velocità normativa. Il Governo, oltre a predisporre risorse per il dissesto idrogeologico, ha previsto strumenti semplificati e di coordinamento tra gli enti territoriali, al fine di raggiungere l'importante obiettivo della sicurezza e della tutela della vita delle persone. Questo è il modo più efficace per esprimere solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime, nonché per confermare l'impegno del Governo e di Fratelli d'Italia a sviluppare strumenti sempre più snelli ed efficaci per la migliore gestione e pianificazione delle politiche in favore del territorio. Richiamare tutti alle loro responsabilità ed evitare sciacallaggi sono le linee del nostro agire. Auspichiamo quindi che anche le Regioni prestino la più celebre attenzione all'aggiornamento dei piani di assetto idrogeologico, così come sarebbe utile un'analisi ricognitiva e valutare l'efficacia degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto adottati dalle Autorità di bacino, al fine di sviluppare la resilienza dell'assetto territoriale in relazione alla numerosità e all'intensità degli episodi alluvionali e franosi nel territorio d'ambito. La tragedia di Ischia pone con drammatica urgenza la necessità di azioni concrete per evitare il dissesto. Nel corso del suo mandato, questo Governo porterà avanti le sue politiche di prevenzione, salvaguardia e tutela dei territori, per la cui buona riuscita sono necessari però anche i seguenti interventi: l'aggiornamento e l'approfondimento continuo dei piani di assetto idrogeologico e gestione delle alluvioni; l'adeguamento della pianificazione urbanistica comunale dei vari Comuni interessati; la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento dei piani di Protezione civile; l'informazione alla cittadinanza e - cosa fondamentale - la manutenzione estensiva del territorio; soprattutto, un piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico. Con questo decreto-legge, il Governo adotta anche misure volte a disciplinare la sospensione dei termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali. All'articolo 4, come ricordava il senatore Rastrelli, viene prevista la proroga al 1° gennaio 2024 per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia, e viene rifinanziato con 10 milioni di euro per l'anno passato il Fondo regionale di protezione civile. civile. Ad onor del vero, grazie alle integrazioni apportate nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, sono stati attribuiti al commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2017 anche i compiti relativi agli interventi riferiti all'alluvione del 26 novembre scorso, al fine di garantire il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili privati. C'è un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso, con i citati 40 milioni per il periodo 2023-2026. Sono incrementate le unità di personale a supporto del commissario per un regolamento straordinario. Infine - e mi avvio alla conclusione voglio esprimere la soddisfazione del Gruppo Fratelli d'Italia per un provvedimento così importante, che supporta il tessuto sociale di una popolazione ferita attraverso azioni di sostegno concreto per le famiglie e per le attività commerciali. Allo stesso tempo, mi sento di impegnare la nostra parte politica a fare tanto altro, tutto ciò che serve e che sarà necessario per l'isola di Ischia e per tutti i territori colpiti da calamità e disastri. Sono anche sicuro che tutti in quest'Aula siano pronti e disponibili a seguire questo percorso. Voglio concludere affermando che, anche se il timore avrà più argomenti, noi sceglieremo sempre la speranza, la speranza che tutto ciò non accada, la speranza che non accada mai più. A tutti i cittadini ischitani voglio dire: abbiate fiducia prima in voi stessi e - se me lo consentono gli onorevoli senatori - abbiate più fiducia in questo Parlamento e in questo Governo, che sono stati vicini ai vostri disagi e lavoreranno ancora per arginare e risolvere le difficoltà che state attraversando. «Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, neppure la notte più buia». Per tutti questi motivi, anticipo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.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

Il Senato tornerà a riunirsi in